in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione

fanno riferimento a integrazioni e previsioni in materia di convenzioni internazionali di rapporto con il nostro codice di procedura penale, in particolare le norme transitorie, quelle di attuazione e coordinamento, per la parte concernente la possibilità di effettuare delle conferenze telefoniche o video conferenze con sistemi audiovisivi,

alle convenzioni internazionali, sia il nostro primo punto di orientamento. Peraltro, siccome in materia abbiamo una competenza e un'esperienza certamente superiori a quelle di molti Stati esteri per quanto riguarda i sistemi audiovisivi e le videoconferenze, riteniamo sia opportuno fare, in parte, rinvio alle norme del codice di procedura penale che già prevedono l'effettuazione delle audizioni, delle trascrizioni e delle registrazioni secondo i meccanismi che ben conosciamo. pare utile fare riferimento soprattutto all'articolo 205-*ter* delle norme di attuazione del codice di procedura penale che prevedono tutte le situazioni, anche per gli imputati, sia nel caso ordinario che possa succedere e, cioè, quello di uno stato di detenzione, ma anche nel caso in cui la persona imputata si trovi - ad esempio - in uno stato di malattia che non ne consente il trasporto. È per questo che va fatto questo riferimento. Se ci fermassimo infatti alle convenzioni internazionali, si lascerebbe al momento uno

l'emendamento 4.202, esso fa riferimento ai poteri del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni richieste in casi particolari per l'esecuzione all'estero o nel territorio dello Stato della sentenza della

specificazione riguarda alla necessità che non esistano contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. L'emendamento 4.203 riferimento a una distinzione che effettuiamo tra sentenze e altre decisioni giudiziarie. Facciamo inoltre riferimento, con una proposta di inserimento, anche relativamente all'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, perché in un caso si parla di Stati dell'Unione europea e, nell'altro caso, di Stati extra Unione europea. È necessario in entrambi i casi che vengano assicurate le garanzie per per le persone, per gli imputati e, in un concetto più ampio, sussumiamo il tutto sotto il concetto e la finalità di garanzia giurisdizionale.

il Parlamento controlla il Governo e il Ministro deve rispondere politicamente delle sue azioni. Noi facciamo invece un sinallagma fra un qualsiasi procuratore della Repubblica e uno Stato sovrano naturalmente i procuratori della Repubblica sono sotto il controllo di nessuno - mettiamo alla pari ogni procuratore della Repubblica con uno Stato sovrano e addirittura gli permettiamo di fare questi accordi anche con Stati al di fuori dell'Unione europea, senza l'autorizzazione del Ministro.

che è stata estradata all'estero: non si capiva bene se la responsabilità fosse del Ministro, del procuratore oppure della polizia. Ne è sorto uno scandalo nazionale, perché si è detto che il Ministro comunque era informato e il capo di gabinetto ha dovuto dimettersi.

una ulteriore conferma di una deriva nella quale il Parlamento abdica a principi fondamentali della democrazia in vigore in tutti i Paesi europei, per delegare funzioni delicatissime, senza alcun controllo politico, a tutti i procuratori della Repubblica insistenti sul territorio. Mi rendo conto che difficilmente questo emendamento verrò accolto, ma è bene che rimanga nella memoria del Parlamento che, mentre c'è tutto un dibattito pubblico sul rapporto tra politica e magistratura, sulla magistratura che fa le leggi e sulla magistratura che si sostituisce al Parlamento, adesso la magistratura assumerà anche poteri che, in tutti i Paesi democratici, sono devoluti all'Esecutivo. E verrà assegnato all'autonomia di ogni procuratore della Repubblica la facoltà di costituire squadre investigatrici comuni con investigatori di altri Paesi. Mi sembra questa una ulteriore strada verso una deriva di confusione tra i poteri dello Stato.

la senatrice Mussini. Se questa proposta aveva un significato, certamente anche politico, quando il testo è arrivato all'esame delle Commissioni riunite successivamente, anche con l'accoglimento di diversi emendamenti (sia della maggioranza che dell'opposizione)

Alla quinta riga, laddove si fa riferimento a «il collegamento audiovisivo», queste parole vengono sostituite con le seguenti: «le varie forme di collegamento a distanza». Alla riga successiva, dove si dice: «condizioni di utilizzabilità tenuto conto di quanto previsto», tra «utilizzabilità» e «tenuto» va inserita la parola «anche»; quindi, la frase diventerebbe: «le condizioni di utilizzabilità anche tenuto conto di quanto previsto».

Per quanto riguarda l'emendamento 4.201, del senatore Giovanardi, faccio presente all'Assemblea che le squadre investigative comuni già esistono, sono uno strumento fondamentale d'indagine per tutta l'Europa e sono state adottate, a seguito di legge del Parlamento italiano proprio due anni fa, con decreti legislativi applicativi da parte del Governo. Sono quindi già funzionanti e riguardano gli Stati dell'Unione europea. Noi ci siamo presi uno scrupolo in più perché, quando si tratta di squadre investigative europee che non fanno riferimento agli Stati dell'Unione europea, il Ministro interviene con la comunicazione dell'accordo formulato, proprio perché sia nella consapevolezza di tutti quanto succede

Grazie

deriva l'opportunità, a rischio di una vistosa sgrammaticatura dal punto di vista costituzionale, della formulazione prevista nell'emendamento Nel nostro ordinamento costituzionale il Ministro della giustizia ha un suo ruolo, non certo per ledere autonomia e indipendenza della magistratura procedente, ma perché, ad esempio, un ruolo di politica internazionale, un ruolo esterno, quindi comunque rapportato in ogni democrazia al controllo parlamentare, passi

Nel caso in cui noi non arrivassimo alla formulazione suggerita nell'emendamento 4.201 e facessimo nostri

in capo a benemeriti procuratori che, fino a prova contraria, sono sì dei magistrati, ma dei funzionari magistrati sui quali il Parlamento

Signor Presidente, richiamo l'attenzione di tutti su questo emendamento, e non solo su questo. I componenti I componenti della Commissione giustizia sanno che su questo provvedimento il nostro Gruppo ha dato un forte contributo muovendosi nella stessa ottica del relatore, con una serie di emendamenti che sono stati accolti o assorbiti proprio perché avevamo la stessa linea interpretativa.

non è una questione politica (mi meraviglierei se per ipotesi dovessimo votare in ragione dell'appartenenza a Gruppi diversi), ma è una ragione istituzionale. Come tutti sapete, in Europa, come quasi in tutto il mondo, il Ministro della giustizia ha il potere

a favore solo del magistrato, che non ha responsabilità politica. Ma noi qui, correttamente, abbiamo introdotto non solo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ma i principi di reciprocità con gli altri Stati.

la necessità di trovare una soluzione e di riflettere, poiché dal Governo (ma non ho capito se dal ministro Orlando o dall'ufficio legislativo del Ministero della giustizia, composto da magistrati) vi era stata un'indicazione contraria a questa soluzione.

diciamo che il Ministro non deve essere nemmeno informato. Ma vi rendete conto che in Francia esiste la discrezionalità dell'azione penale e la dipendenza dal Ministro della giustizia? E che anche in Germania, dove c'è

Grazie prima di votare l'emendamento, non solo ci sia una riflessione, ma che il relatore, nel quale confido, intervenga sul Governo - e non solo su questo

Il collega Caliendo giustamente ha sottolineato che degli accordi che intervengono tra procuratori e Stati sovrani europei il Ministro della giustizia non ne sa assolutamente nulla perché non gli deve essere notificato nulla e già questa è un'anomalia gigantesca, ma nel caso di Paesi non europei il testo che

Vi sembra possibile che si costruisca un sinallagma di questo tipo, che è una frattura costituzionale gigantesca? Da quando i procuratori della Repubblica possono fare, ognuno di loro, politica internazionale e stabilire di fare squadre di investigazione comune anche sul nostro territorio, senza alcun controllo

Signor Presidente, chiederei al relatore una riformulazione che limiti questa autonomia soltanto ed esclusivamente ai Paesi appartenenti all'Unione europea

non sono squadre operative, ma squadre investigative comuni previste dal diritto internazionale europeo e dallo Stato italiano. Cito in particolare, per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, la decisione quadro del 13 giugno del 2002. A seguito di quella decisione, che risale ormai a quattordici anni fa, si doveva procedere all'approvazione di norme del nostro diritto interno per la formazione e la previsione di queste squadre investigative comuni, secondo le indicazioni che venivano da questa decisione quadro.

ha imposto agli Stati membri di adottare questo strumento investigativo comune all'interno degli Stati facenti parte dell'Unione europea. Allo stato attuale, fin dall'anno scorso, tutti gli Stati dell'Unione europea avevano adottato questo strumento investigativo; l'ultimo rimasto era lo Stato italiano, che non aveva provveduto. In questa legislatura c'è stato un intervento normativo da parte del Parlamento (da ultimo, in particolare, un decreto legislativo del 15 febbraio 2016, quindi passato ovviamente attraverso le Commissioni parlamentari per quanto di competenza, che adottava anche per l'Italia lo strumento delle squadre investigative comuni, con particolare riferimento a tutta una serie di reati gravissimi, quali la lotta al terrorismo e alla grande criminalità organizzata. Ricordiamo tutti - anche il Popolo della Libertà con cui abbiamo lavorato in Commissione - che c'è stata una segnalazione all'inizio di quest'anno, proprio a seguito dei gravi fatti criminali terroristici,

Grazie

Questa indicazione veniva ribadita dal Governo e da questo disegno di legge in prima battuta. Come Commissioni giustizia ed affari esteri del Senato ci siamo fatti carico di questo tema e abbiamo previsto un di più, nel senso che di questo deve essere data comunicazione al Ministro della giustizia quando si tratta di formulazioni e di accordi con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, ovviamente per quanto di competenza del Ministro. questa comunicazione, scritta nel rispetto del diritto europeo e del diritto internazionale. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione l'intervento del relatore Casson. Qui non è in discussione la costituzione e l'operatività delle squadre investigative comuni, ma quale autorità il potere di interloquire in ordine a tale costituzione. Secondo il concetto espresso dal senatore Casson, capo all'autorità giudiziaria, che può sostanzialmente prendere accordi con corrispondenti autorità di altri Stati per tale costituzione. Giustamente il senatore Caliendo, poco fa, ha fatto notare all'Assemblea come questa formulazione consentirebbe in astratto ad uno dei 126 - se non ricordo male - procuratori della Repubblica esistenti in Italia di prendere, ad esempio, un accordo diretto con il Ministro della giustizia americano, essendo evidentemente l'*Attorney general*, cioè il Ministro della giustizia americano, l'autorità competente alle squadre investigative comuni.

siccome si parla di Stati diversi dall'Unione europea, apro e chiudo una parentesi: il Ministro della giustizia francese può bloccare la costituzione delle squadre investigative comuni in ragione del diritto interno attuativo delle convenzioni cui faceva il riferimento il senatore cui faceva il riferimento il senatore Casson. Il problema allora è questo; se la costituzione delle squadre investigative comuni, per qualsivoglia ragione, non necessariamente nota al sopra citato procuratore della Repubblica di Larino, può mettere in dubbio e in crisi le esigenze di sicurezza nazionale, può l'autorità di Governo in qualche modo interloquire? Questa possibilità di interlocuzione - che mi sembra ispirata esclusivamente al buonsenso - può essere soddisfatta con la mera comunicazione? A che serve, senatore Casson, dare comunicazione al Ministro della giustizia, se poi non si prevede, in ragione di questa comunicazione, una possibilità di intervento di quest'ultimo? quest'ultimo? Siccome viviamo in questo Paese e sappiamo bene che il Ministro della giustizia difficilmente negherà un'autorizzazione, ove questo diniego dovesse essere strumentale a ragioni non solide, credo allora che affermare, come si fa nell'emendamento 4.201, «previa autorizzazione del Ministro della giustizia», a mio avviso renderebbe la norma sicuramente operativa, ma sicuramente più consona a quelli che sono i principi generali del nostro ordinamento, richiamati poco fa dal senatore Compagna. In altri termini, si chiede che in condizioni di assoluta reciprocità con altri Paesi, ivi compresi quelli dell'Unione europea (perché la Francia, come ricordavo prima, consente al Ministro della giustizia di bloccare le squadre investigative comuni), si proceda alla costituzione delle squadre investigative comuni anche il procuratore della Repubblica di Larino possa, in ipotesi, costituire con il Ministro della giustizia americano queste squadre investigative comuni), a condizione però che il Ministro della giustizia italiano sia previamente sia previamente reso edotto di quanto sta accadendo e autorizzi, com'è normale che sia, tale costituzione. Questo è in estrema sintesi il problema.

insomma, nel momento in cui questa costituzione di squadre investigative comuni dovesse essere posta in essere con problemi rilevanti per la sicurezza di questo Paese, secondo voi ne risponderà il procuratore di Larino o il Ministro della giustizia? Davvero voi ritenete che su un sistema così delicato il Governo e il Ministro della giustizia debbano adottare la politica dello struzzo, mettendo la testa sotto terra, per poi difendersi, ove mai dovesse accadere qualcosa, dicendo che in fin dei conti non ne sapevano nulla e che la comunicazione gli è stata

dai relatori. Vengo ora al contenuto. Il disegno di legge che abbiamo oggi all'esame del Senato muove dell'assunto, chiarito nella sua originaria relazione introduttiva, della inadeguatezza dell'attuale sistema normativo di assistenza giudiziaria, a fronte di una criminalità, specialmente quella organizzata, che ha esteso il proprio raggio di azione ben oltre i confini del territorio di un singolo Stato e che sa ben sfruttare tutte le opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati e delle nuove tecnologie di comunicazione e di gestione dell'informazione. Il testo, operando su diversi piani di intervento consistenti nella ratifica di Accordi internazionali, in una proposta di delega legislativa nonché in un diretto intervento di modifica su alcune norme del codice di procedura penale, riguarda la materia della cooperazione ed assistenza giudiziaria per il contrasto dei fenomeni criminali. Il proficuo lavoro svolto in Commissione ha fatto sì che gli aspetti di criticità e di distonia normativa presenti nel testo licenziato dalla Camera possano ritenersi superati anche grazie all'apporto delle proposte emendative che, come Gruppo dei Conservatori e Riformisti, abbiamo portato in sede di Commissione e che i relatori, in molti casi, hanno fatto propri. Mi preme, in particolare, sottolineare come il testo che stiamo votando abbia recepito le nostre istanze circa il necessario rispetto del fondamentale principio di reciprocità nelle domande di assistenza giudiziaria e di estradizione, con particolare riguardo ai Paesi extra-UE, ove tale condizione od analoghe garanzie possono non essere disciplinati da atti pattizi internazionali. Così come ritengo positivo il recepimento di un altro nostro emendamento finalizzato a fissare dei precisi parametri in base ai quali l'autorità giudiziaria competente deciderà se accogliere o no la richiesta di assistenza giudiziaria. Tali criteri sono quelli forniti dall'articolo 724, quinto comma, del codice di procedura penale, per il diniego di esecuzione delle rogatorie con riferimento alla compatibilità della richiesta di assistenza con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con la legge penale all'assenza di pregiudizi persecutori nei confronti dell'imputato che non abbia prestato il proprio consenso. Concludo con la modifica apportata alla novella in tema di estradizione ove, nel rispetto dei principi fondanti il nostro ordinamento giuridico, è stato inserito il principio della doppia imputabilità, in forza della quale non si può essere estradati per qualcosa che nel nostro Paese non costituisce illecito penale. Ciò eviterà che le persone possano ritrovarsi accusate di reati di cui non conoscevano neppure l'esistenza perché molte condotte - tra le quali, i cosiddetti reati d'opinione - possono essere valutati in modo diverso nelle varie giurisdizioni. In forza di queste considerazioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo dei Conservatori e Riformisti al provvedimento in esame.

Si tratta di passaggi necessari, affinché si possa creare una vera barriera contro la criminalità.

importante che tutti gli Stati collaborino e il principio di reciprocità sia uno stimolo affinché venga attuata una collaborazione vera, che non deve mai essere solo unilaterale.

È per questo che noi voteremo sempre i provvedimenti che comportano una vera e seria lotta contro la delinquenza e voteremo sempre contro tutti quei provvedimenti che invece comporteranno dei benefici

Ma, signori, se non si è uno Stato serio sotto il profilo della giustizia, se la giustizia non è credibile, uno Stato diventa non più credibile.

è espressione di un Governo in carica ed è espressione proprio di quella parte del Parlamento che ha bocciato l'emendamento. Certo che c'è un problema politico di fondo. Il presidente Renzi è venuto qua a raccontarci, l'altro giorno, tutta una serie di belle cose rispetto alla giustizia, ma la realtà è sotto agli occhi di tutti: la politica giudiziaria della maggioranza, del Governo e del PD, gloria PD, gloria loro, la fanno i colleghi Casson e Lumia. È chiaro che il Governo è a trazione Casson-Lumia. Il prodotto legislativo che esce dalla Commissione giustizia e dal Parlamento, dall'omicidio stradale stradale al disastro ambientale, fino al discorso della prescrizione, è esattamente il rovescio di quello che ci viene a raccontare il Presidente del Consiglio. È evidente che si tratta di un problema di fondo, che arriva perfino a scavalcare il Parlamento e il potere esecutivo, pur di dare più potere ai magistrati, come la votazione di oggi ha dimostrato. Per questi motivi, pur condividendo larga parte del contenuto di questo disegno di legge, noi ci esprimiamo per l'astensione.

Signor Presidente, dirò poche parole per annunciare il nostro voto a favore della ratifica in esame. Ovviamente anche noi condividiamo le parole di chi ha detto che la ratifica arriva con molti anni di voto sarà favorevole perché la Convenzione risponde alla necessità di migliorare la cooperazione giudiziaria, senza pregiudicare però le norme che tutelano la libertà e soprattutto continuando ad assicurare l'assistenza giudiziaria in maniera rapida ed efficace, compatibile con i principi fondamentali del diritto interno dei singoli Stati appartenenti all'Unione europea, nel rispetto dei diritti individuali. La mancata ratifica, in tutti questi anni, della Convenzione da parte dell'Italia ha ovviamente contribuito a delegittimare ed indebolire il nostro Paese nelle organizzazioni internazionali, ma ha anche impedito, ad esempio, un lavoro che poteva essere fatto per ricostruire la verità e per garantire giustizia alle vittime della strage di Ustica. Proprio in assenza della ratifica di questa Convenzione, nel Parlamento europeo non è stato possibile per l'Italia chiedere una cooperazione che potesse riportare verità su quei fatti. Noi voteremo dunque a favore, nonostante non abbiamo condiviso l'inserimento alla Camera della delega al Governo per riformare il libro XI del codice di procedura penale e la modifica di alcune disposizioni in materia di estradizione

proprio per limitare, dando indicazioni più precise, una delle ennesime deleghe che questo Governo tenta tutte le volte di riservare a sé. Lo vogliamo ribadire, perché ogni volta che si conferisce una delega troppo ampia al Governo si continua

relativa all'assistenza giudiziaria del 29 maggio 2000, già operativa, con ratifiche interne, in 24 Paesi dell'Europa,

Dove e come si è mossa la Convenzione sull'assistenza giudiziaria del 2000? Si è mossa su un quadro normativo costituito dalla Convenzione europea del 1959,

Bisogna dare atto al relatore e al Governo che in Commissione c'è stata una discussione approfondita, che ha visto una disponibilità al ragionamento per portare all'emanazione di un provvedimento che fosse il più corretto possibile. Molti sono stati gli emendamenti

dubbio interpretativo che questa mattina, al di là del voto favorevole dichiarato da tutte le forze politiche, ha dato adito a qualche discussione interna.

sono norme primarie, alle quali il diritto interno si deve attenere. È, ovviamente, la classica graduazione della classificazione delle norme tra norme primarie e norme secondarie. la norma interna è norma secondaria rispetto alla norma primaria. Quindi, probabilmente, tralasciando questa visione ampia del sistema normativo di riferimento, il senatore Compagna si è lasciato andare addirittura a qualche rilievo di incostituzionalità del provvedimento di legge che stiamo oggi approvando. Altro rilievo devo fare al senatore Palma. È nota la mia ammirazione per la maestosa preparazione del senatore Palma.

con il Presidente degli Stati Uniti d'America la costituzione di una squadra investigativa comune. Ci sono dei passaggi che tale procuratore deve fare

sia per la crisi economica sia per il fenomeno del terrorismo, tutte le forze politiche all'interno di ogni Stato europeo (e non solo) devono collaborare per arrivare all'obiettivo di sconfiggere questi cancri che vengono dall'esterno a distruggere le nostre società. esame è uno strumento importante e devo dare atto a tutte le forze politiche (Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Conservatori e Riformisti,

momento in altri Paesi europei vediamo Governi di unità nazionale, auspico che non solo sul provvedimento in esame, ma su tutti quelli che andremo ancora ad adottare ci possa essere una visione di unità nazionale

chi va dal Presidente della Repubblica ad eccepire violazioni di norme costituzionali tralasciando di considerare che il principio generale primario della nostra Costituzione è l'autonomia del mandato

all'assistenza giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell'Unione europea. Molti dei colleghi hanno già rappresentato degnamente le ragioni di questo assenso; ne ripercorro molto brevemente i tratti salienti e poi farò una considerazione puntuale su un emendamento in particolare che è stato respinto e che avrebbe potuto essere valutato, soprattutto dal Governo, in maniera diversa. Perché siamo a favore di questa ratifica? Non solo per uniformità e coerenza con quanto è stato definito in sede europea (organismo, l'Unione europea, di cui siamo Paese fondatore e primari protagonisti della sua funzione), ma anche e soprattutto perché questa ratifica consente al nostro sistema giudiziario di poter svolgere più tempestivamente e con maggior incisività i compiti di istituzionali propri attraverso la semplificazione e la maggior efficacia delle formalità di procedure che sono inerenti all'assistenza giudiziaria con gli altri Stati membri. Si introducono anche forme tecniche specifiche per rafforzare questa possibilità di collaborazione e, insieme a questa ratifica, vengono conferite al Governo alcune deleghe per la riforma del libro XI, che concerne

l'intervento che facciamo è cautelativo della qualità di uomo libero anche della persona sottoposta a indagini, che può essere evidentemente compromessa e attenuata da misure che, nell'interesse collettivo alla tutela della sicurezza pubblica, hanno una prevalenza rispetto al bene della libertà personale. C'è un'accentuata esigenza di collaborazione internazionale che si sposa con l'amplificata pericolosità del crimine, non solo per finalità economiche, ma anche per obiettivi dichiarati di aggressione all'intero sistema istituzionale del mondo libero e dell'Occidente in particolare. Per tali finalità, è quanto mai opportuno che questa collaborazione avvenga in maniera appropriata con sveltimento dei procedimenti e con la costruzione di un sistema giudiziario moderno che consenta al nostro Paese di adeguare il proprio ordinamento rispettando sia la lotta alla criminalità sia la tutela dei diritti fondamentali del cittadino, che mai vorremmo fossero sacrificati ad altri argomenti. C'è un unanime riconoscimento, nelle motivazioni di questo provvedimento, per una qualificata inadeguatezza di alcune procedure, di alcuni meccanismi del nostro sistema che hanno anche fondamento normativo, che denotano un'eccessiva laboriosità di una prassi applicativa Il punto su cui esprimo un'opinione critica

lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità o in caso di pericolo per la sovranità e la sicurezza degli interessi nazionali dello Stato, argomento quanto mai condivisibile. E qui esprimo, forse a titolo personale, un punto di vista differente da quello del Governo sul tema specifico che riguardava l'emendamento che considerava ininfluente la volontà del Ministro, che era soltanto oggetto di informativa, per la costituzione di squadre investigative comuni

comunicato, espresso ed assodato sui valori di fondo e sulla necessità ed opportunità di varare questa iniziativa, su questo punto abbiamo rinunciato

membri delle Forze dell'ordine di Stati stranieri sul nostro territorio delle funzioni investigative e altro, questo possa avvenire solo ed esclusivamente con l'avallo consapevole e circostanziato dell'Esecutivo. Se i relatori possono avere un'opinione diversa, mi meraviglia che il Governo abbia rinunciato esso stesso ad affermare una prerogativa che fa parte delle funzioni istituzionali del Governo medesimo.

alla correzione del testo pervenuto dalla Camera dei deputati. La correzione non è stata indotta da logiche di Gruppo o politiche, ma da un'attenta considerazione di alcuni principi fondamentali e devo riscontrare una condivisione con il relatore Casson e con il Governo delle modifiche

nel nostro Paese il Ministro si è sempre adeguato e non ha mai contraddetto le richieste della magistratura. Mi domando, quale sia la ragione per cui oggi andiamo a sminuire ulteriormente il nostro Paese nei rapporti con gli altri Paesi. Il relatore Casson e gli altri sanno meglio di me che i ritardi, in una effettiva procura europea, dipendono proprio dalla diversa posizione dei vari Paesi. Da noi vi è la concezione che il potere giudiziario è solo nelle mani dei magistrati, anche se si dovrebbero ogni tanto leggere i verbali dell'Assemblea costituente per rendersi conto di quali erano i valori che in quella sede venivano indicati.

alla soluzione italiana perché furono introdotti i membri laici del Consiglio superiore della magistratura, pensando in tal modo di poter determinare un equilibrio.

il nostro Paese è riconosciuto all'estero come portatore di forti indicazioni dal punto di vista tecnico-giuridico, ma non è considerato per l'incapacità di esprimere, sul piano politico e a livello generale, una posizione che sia rappresentativa, anche in relazione alle cariche rivestite, di una forte istituzione Paese.

vuol dire che le stesse iniziative dei procuratori della Repubblica avranno un minor peso nel momento in cui si troveranno a dialogare con Ministri di altri Paesi che hanno un potere effettivo, di responsabilità politica. I nostri pubblici ministeri hanno potere giudiziario all'interno, ma non hanno responsabilità politica, non impegnano il nostro Paese su alcune scelte e quando vi è da valutare l'interesse dello Stato

(mi auguro) ad un'azione di convinzione morale del procuratore della Repubblica, ove si muova in una direzione sbagliata. Queste sono le ragioni per cui noi,

l'inefficienza del nostro sistema parlamentare: non vi è la capacità di discutere su questioni che non attengono a scelte politiche dei rispettivi Gruppi, prescindendo dalla disciplina di Gruppo. Se si vuole Gruppo. Se si vuole ragionare in termini di una legislazione efficiente, specialmente quando non sono in forse programmi, ideologie proposte di ciascun partito, si deve avere la capacità di astrarsi dallo schieramento di Gruppo e individuare piuttosto soluzioni

Presidente, colleghi, ci troviamo di fronte ad un atto che il Parlamento ed il Senato approvano dopo anni e anni di attesa. Ricordo a tutti i colleghi che siamo fermi ad una Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio del 2000. Il nostro Paese in queste settimane, in questi mesi, si sta battendo in Europa per fare in modo che nella lotta al terrorismo si possa finalmente procedere in un'ottica integrata integrata e comune e non più in un'ottica di semplice cooperazione, perché nella pur positiva cooperazione non riusciamo

aspetta 16 anni per dar vita alla richiamata Convenzione del 2000? Capite che c'è una contraddizione che finalmente sciogliamo positivamente. Adesso il nostro Paese potrà dire di avere le carte in regola per battere i pugni sul tavolo e fare in modo che a livello europeo non solo si armonizzino tutte le legislazioni (e noi siamo ben ultimi a fare questo lavoro),

ad un coordinamento europeo e ad uno spazio giuridico antiterrorismo e antimafia comune, che preveda addirittura la procura europea antimafia e antiterrorismo. Ecco qual è la meta, l'obiettivo e la visione che dobbiamo avere in questi secondi e in questi minuti, in cui ci accingiamo a votare questo importante provvedimento. Cari colleghi, ricordo a tutti che l'articolo 117 della Costituzione recita «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,» come è ovvio, «nonché» ed ecco il punto «dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Quindi, cari colleghi, non ci siamo mossi al di fuori dei vincoli che noi abbiamo. Anzi, ringrazio quanto fatto dalla maggioranza e dall'opposizione nelle due Commissioni, giustizia ed affari perché siamo riusciti a fare un lavoro di cesello delicatissimo affinché la nostra storia e le nostre garanzie non venissero meno. Un lavoro molto complesso, ma penso, alla fine, ben riuscito. Ecco perché, colleghi, ci apprestiamo a fare questo passo in avanti. È un passo in avanti che, come la senatrice Ginetti nel suo intervento ha saputo ben spiegare, tiene conto di un più complesso lavoro che si è fatto sulle direttive europee che riguardano diversi elementi che vanno ad integrare quello che stiamo facendo adesso. Alla fine, potremo dire che questo Paese ha le carte in regola perché l'Europa abbia finalmente uno spazio giuridico antiterrorismo, antimafia, antidroga e antitratta comune e può procedere,

«è quello di analizzare il legame tra le attività, la gestione e la situazione economico‑finanziario di ENI SpA e delle società interamente partecipate o controllate dalla stessa e il fenomeno della corruzione, che presenta per la sua dimensione, estensione e profondità, connessioni dirette con il sistema politico, con la pubblica amministrazione, con il sistema delle autonomie locali, con i corpi tecnici e con i funzionari dello Stato, con il mondo delle imprese e più in generale dell'economia e della finanza.». Infatti, signor Presidente, «ENI è stata ed è a tutt'oggi parte in numerosi procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegati allo svolgimento delle attività industriali, nonché in diversi contenziosi fiscali». Di questi, citerò solo i principali: principali: dal contenzioso relativo all'omesso pagamento ICI per alcune piattaforme petrolifere localizzate nelle acque territoriali del Mare Adriatico, all'accertamento per la concessione di Cabinda in Angola; vi sono poi i procedimenti relativi alla raffineria di Gela, i procedimenti relativi alle aree site nei Comuni di Cassano allo Ionio e Cerchiara di Calabria, le indagini che interessano la Syndial SpA nel sito di Crotone e il processo che vede imputate la Syndial e la Versalis SpA, questa volta per disastro ambientale, nel Comune di Porto Torres. Ma quello che desta grave preoccupazione, a mio modo di vedere, sono i presunti casi di corruzione e, segnatamente, di corruzione internazionale. Infatti, ci sono ipotesi di corruzione internazionale relativi all'attività di ENI in Kazakhstan, un parallelo filone di indagine che la coinvolge in attività condotte in Iraq ipotesi di reato di corruzione internazionale che coinvolgono ENI e il gruppo Saipem, da essa controllato, in Algeria. Per finire, caso di cui si è occupata tutta la stampa nazionale e internazionale, un'ipotesi di corruzione internazionale per ottenere la concessione decennale nel campo di esplorazione petrolifero denominato Opl-245 al largo della Nigeria. Con questa richiesta di procedimento d'urgenza vorrei sottolineare che io, a nome del Gruppo Movimento 5 Stelle, reputo necessario ed urgente approfondire soprattutto le ragioni che hanno portato a tali operazioni nonché comprendere quali correttivi possano essere apportati a livello normativo per rendere più trasparente la gestione della società che ha una partecipazione pubblica e per contrastare più efficacemente la corruzione. A tale proposito ricordo le parole che il presidente Mattarella ha detto proprio ieri ai Capigruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato che lo hanno incontrato, parole che ricordano, ancora una volta, quanto sia alta l'attenzione della Presidenza della Repubblica riguardo ai numerosi casi di corruzione che coinvolgono la pubblica amministrazione, ma anche le imprese italiane, e io direi proprio in questo caso, una grande impresa a partecipazione pubblica. Poiché le indagini della magistratura, ma non solo, che chiamano in causa dirigenti di rilievo del gruppo e anche persone collegate alla dirigenza, esigono che si faccia la massima chiarezza, tenuto conto che tali fatti si scontrano con gli obiettivi che ENI proclama di perseguire nella lotta alla corruzione, io penso che, a parole, l'azienda debba continuare con questa filosofia, ma nei fatti debba assolutamente mettere in pratica quanto ha scritto nel proprio codice etico. Infatti, nel codice etico di ENI sono vietate espressamente «pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi,

per prevenire e contrastare atti di corruzione, a me sembra evidente che il coinvolgimento del *management* di ENI, nei diversi e presunti casi che ho già citato, susciti forti dubbi in merito alla reale efficacia degli standard etici e anticorruzione di cui le società in generale si dotano e, in particolare, del ruolo che ai fini anticorruttivi e di illegalità può svolgere l'azionista pubblico nelle società a partecipazione statale, e sottolineo l'azionista pubblico. Per questi motivi il mio Gruppo parlamentare propone l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta. questa proposta è totalmente scollegata dai fatti di cronaca di cui abbiamo anche parlato nel corso della discussione sulla mozione di sfiducia al Governo, discussa proprio in questi giorni qui al Senato, ma so e sappiamo che alla Camera dei deputati è stata presentata una Commissione parlamentare d'inchiesta monocamerale che però è fortemente centrata sulle questioni di cronaca. A seguito delle parole del presidente della Repubblica Mattarella e a seguito delle vicende che stanno coinvolgendo, e non dovrebbero coinvolgere,

non debba in alcun modo interferire con esse, lasciando alla magistratura l'esercizio pieno e libero delle sue funzioni e delle sue attribuzioni. Stiamo inoltre parlando di una grandissima multinazionale italiana, forse l'unica grande multinazionale che è rimasta al nostro Paese: una società quotata in borsa, che ha grandi responsabilità, non soltanto nei confronti delle decine e decine di migliaia di lavoratori che che ha in corso trattative internazionali per l'utilizzo di risorse energetiche, di cui il nostro Paese ha una Si tratta di una società alla quale l'Italia deve garantire naturalmente la massima stabilità e le massime

in questo processo, anche soltanto con l'annuncio di un dibattito su possibili inchieste parlamentari francamente mi sembra improvvido, da un punto di vista istituzionale, politico e anche con riguardo alle strategie del

Non siamo in corso di votazione, senatore D'Anna.

(anche del passato, com'è noto), che ci sia la possibilità di dar vita in modo rapido (con il dimezzamento dei tempi, così come prevede l'articolo 77) a questa Commissione di inchiesta.

tutto alla magistratura, le cui indagini faranno il proprio corso senza che vi sia assolutamente alcuna possibilità di interferenza o di sovrapposizione. questo serva proprio per l'assunzione di responsabilità politiche, per far luce sulle responsabilità politiche e per far luce anche su come agisce, nel caso specifico, una grande società

(se ci sono stati, ovviamente e questo la Commissione di inchiesta dovrà appurarlo), che invece hanno fatto in modo che la società si trovasse - come purtroppo è emerso anche dai recenti fatti - implicata in comportamenti che danneggiano l'interesse pubblico, l'interesse collettivo e, nel caso specifico dell'inchiesta di Potenza e della Basilicata, la salute pubblica. Quindi, a maggior ragione, noi voteremo a favore. Presidente, premesso che certamente creare una Commissione di inchiesta è legittimo, perché è previsto dai nostri Regolamenti, faccio notare che l'ENI è una società quotata in borsa,

perché il Parlamento abbia cognizione di alcuni aspetti peculiari. Ma francamente una Commissione di inchiesta non mi sembra appropriata. Signor Presidente, il Gruppo di Area Popolare voterà contro questa proposta, per due motivi. Il primo motivo riguarda la Commissione di inchiesta in quanto tale. Noi non siamo in assoluto contrari alle Commissioni d'inchiesta. Come ricordava il senatore Carraro, sono previste e ne sono state istituite tante nel Parlamento italiano. Riteniamo, però, che la Commissione d'inchiesta in quanto tale sia un evento straordinario; non un fatto di non un fatto di *routine*, non un disegno di legge approvato di *routine*. E siamo ancora più convinti dell'eccezionalità di una Commissione d'inchiesta agli scarsi esiti che hanno avuto tutte le precedenti Commissioni d'inchiesta istituite, in modo congiunto da Camera e Senato o dal solo Senato:

stati portati all'evidenza pubblica da indagini giudiziarie. Ed è giusto, anzi ci sembra assolutamente necessario, che proprio l'autorità giudiziaria accerti e concluda le indagini, che almeno concluda una buona parte dell'indagine e del processo penale o civile, senza interferenze e senza sovrapposizioni.

assoluta contrarietà a fare delle Commissioni d'inchiesta un oggetto di polemica politica. Per questo motivo confermo il voto contrario del nostro Gruppo. Signor Presidente, è di tutta evidenza che la proposta dei colleghi del Movimento 5 Stelle di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sull'ENI è del tutto strumentale. Noi, come Gruppo Autonomie, non condividiamo l'ipotesi perché sarebbe un doppione inutile, con il ruolo e le funzioni sostanzialmente concorrenti con le inchieste poste in essere dalla magistratura. Chiedere al Senato di istituire una commissione monocamerale sulla base di presunti fenomeni corruttivi, allo stato non accertati e giudicati in sede giudiziaria, e di presunte responsabilità penali e civili dell'ENI in relazione alle sue attività industriali, appare come una dichiarazione di sfiducia nei confronti dell'azione della magistratura. Le finalità che sarebbero attribuite alla Commissione, sulla base della proposta del Gruppo del Movimento 5 Stelle, sono, a nostro giudizio, illegittime sotto alcuni profili e ultronee sotto altri. Nella proposta di istituzione della Commissione si afferma di voler indagare sui fenomeni corruttivi che sarebbero emersi e, nel contempo, di verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti. L'accertamento di fenomeni illeciti può essere motivato dall'esigenza di attribuire alla Commissione poteri di inchiesta perché - si ritiene - non esaustivi e probanti l'azione e il giudizio in sede giudiziaria. È una delle ipotesi possibili che tuttavia, a nostro giudizio, decade o, al contrario, diventa pericolosa, se ciò avviene quando si deve attendere l'esito dell'attività di indagine della magistratura in ordine a queste gravi ipotesi di reato e di corruzione. Ebbene, nel caso che ci occupa la magistratura sta esercitando i propri poteri e non ha affatto rinunciato al proprio ruolo. Pertanto, non c'è alcuna necessità di questa Commissione d'inchiesta. Sotto altro profilo è evidente che

In altri termini quest'Assemblea si è già pronunciata sotto il profilo politico e parlamentare, ha ritenuto necessarie e opportune le dimissioni dell'ex ministro Guidi ai fini della piena integrità dell'azione e del ruolo del Governo,

in questo modo ad una profonda distorsione della natura delle Commissioni di inchiesta parlamentare, che in primo luogo sono state concepite come un istituto di garanzia per le opposizioni: distorsione e strumentalità che consideriamo infatti irresponsabili. Per queste ragioni e poiché

e la separazione dei poteri. Tuttavia, proprio nell'attività parlamentare ormai da parecchie legislature noi abbiamo dato vita e diamo vita ogni volta al principio di legislatura, a quell'autentico mostro (in senso antitetico ai principi richiamati) della Commissione antimafia: sempre la stessa, sempre con le stesse prerogative e ormai diventata luogo non capisco se di collaborazione con il Ministro dell'interno nello scioglimento di questo o quel Comune, di esibizione di liste pulite o di liste sporche in occasione delle elezioni comunali. Da questo punto di vista,

troppo specifica, troppo motivata sulla recente vicenda che coinvolge alcuni protagonismi. Invece, nel nostro Gruppo, proprio sulla base di quella vicenda, ma con l'assoluta garanzia dei profili costituzionali, ci sembrava che la proposta del collega Di Maggio, non ancora giunta all'attenzione dell'Assemblea, non presentasse

dalla metà degli anni Sessanta (primo presidente l'onorevole Amadei), la Commissione antimafia è sempre stata bocciata ogni volta che la si è voluta costituire dandole un orientamento, per esaminare il pentitismo: ricordo un disegno di legge dell'ex capo dello Stato Cossiga, che avevamo firmato in circa senatori. La Commissione antimafia è una specie di Commissione permanente, di Commissione d'inchiesta le cui prerogative non sono riuscite neanche a tenere il passo della legislazione antimafia: che c'è lo scioglimento dei consigli comunali, noi abbiamo ancora questo stranissimo rituale della Commissione antimafia. Da questo punto di vista, essendo pregiudizialmente favorevole a un'ampia revisione dei poteri d'inchiesta, ma attraverso una

Carraro sulla formulazione della Commissione dei colleghi del Movimento 5 Stelle, che potrebbe essere svolta come indagine conoscitiva in altra sede. Ma ci riserviamo invece di sostenere, nel più ampio spettro della specificità dei profili politici, non giudiziari, della questione lucana,

per un atto di grande responsabilità, soprattutto anche di saggezza, perché ENI è una parte molto importante della realtà economica del nostro Paese. Ma non vorrei far passare il messaggio che coloro i quali non vogliono la Commissione d'inchiesta sono coloro che vogliono insabbiare tutto. Questo messaggio non può passare. Io ritengo che ci siano organismi di controllo ed organismi terzi che, in ogni caso, se mai ci fosse stato qualche reato o qualche altro problema all'interno dell'ENI, sono deputati

Ora c'è stato un accordo con la Provincia autonoma di Trento per cui questa autostrada non si farà e, tuttavia, la società sembra dare

ha regalato 1.200 milioni, che sono dei cittadini italiani, a una società privata. Il Governo dovrebbe avere la decenza di rispondere. La vendita sembra che sia fissata per la giornata di domani. Spero che il Governo risponda o si occupi del problema.

Signor Presidente, gradirei che i colleghi del Movimento 5 Stelle, prima di andare via come cavallette come hanno fatto ieri... PRESIDENTE. Senatrice Bencini, lei si rivolga alla Presidenza perché qui non stiamo a fare questioni

e all'emozione (oltre che alla fortuna) di potersi esprimere in quest'Aula. Ecco perché ci scriviamo i discorsi, per cercare di essere chiari, concisi e non perdere il filo,

Il punto è che questo video è stato postato da Nicola Virzì, membro dello *staff* comunicazione del Movimento 5 Stelle, assunto e pagato dal Gruppo con i soldi del Senato. Quindi, si tratta di soldi pubblici di tutti coloro che pagano le tasse. Il video, postato su un *social*, sulla pagina del signor Nicola Virzì, "Nick il Nero", è stato fatto a scopo denigratorio, affinché io fossi esposta al cosiddetto pubblico ludibrio in quanto ci sono commenti volgari e violenti, oltre al fatto che ha avuto 106 condivisioni. Ora, sono veramente stufa di questa modalità di fare comunicazione politica. Capisco che il signor Virzì ("Nick il Nero") sia, diciamo, un *server* della Casaleggio *&* co. e del Movimento 5 Stelle; di fatto non credo sia più tollerabile né accettabile tale modalità di screditare l'avversario politico, le persone, per accreditarsi consensi e *click*. Questa modalità rappresenta la nefandezza di questo partito politico, un partito di incapaci, di inetti. La loro produttività è dovuta tutta al loro gruppo legislativo altamente preparato e laborioso:

Colleghi, un conto è il fatto personale, altro è screditare dei colleghi sfruttando il fatto personale. Si riallinei ad un linguaggio più consono all'Aula, altrimenti non accetto provocazioni qui dentro. mi riallineo ad un linguaggio più consono all'Aula. Ha veramente ragione, Presidente, mi scuso e mi dispiaccio, mi dolgo anche e mi pento. Oramai comunque sono tre anni che questi cittadini portavoce

Grazie